Questa mattina si svolgerà la discussione sulla seconda relazione della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Le votazioni sulle proposte di risoluzione avranno luogo oggi pomeriggio. Seguirà nella seduta pomeridiana di oggi - in luogo del sindacato ispettivo, rinviato al pomeriggio di giovedì 20 gennaio - la discussione di mozioni sulla persecuzione dei cristiani.

La prossima settimana, nella giornata di martedì 18 gennaio si terranno due sedute: nella seduta antimeridiana, dalle ore 11 alle ore 13, saranno discusse mozioni sull'estradizione di Cesare Battisti; nella seduta pomeridiana, a partire dalle ore 16, si svolgerà il dibattito sulla relazione annuale concernente l'amministrazione della giustizia. In tale ambito è stato richiesto che il Ministro della giustizia riferisca anche sulla questione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari. A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 19 gennaio, sarà esaminato il decreto-legge sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, già approvato dalla Camera dei deputati.

che sicuramente coinvolgono tutti noi, interessano tutti gli italiani e che, altrettanto sicuramente, ognuno di noi vorrebbe definitivamente

la relazione sul secondo anno di attività della Commissione appare opportuno formulare alcune riflessioni e proposte per segnalare le principali questioni ancora aperte in materia di salute e sicurezza del lavoro sulle quali la Commissione ritiene opportuno richiamare l'attenzione e gli sforzi dei vari soggetti competenti, pubblici e privati, nonché per tracciare le direttrici lungo cui essa intende continuare la sua inchiesta. La prima esigenza fondamentale è ancora una volta quella di assicurare il completamento in tempi rapidi dell'attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche alla luce delle successive modifiche ed integrazioni. Il punto essenziale è quello di procedere all'adozione dei vari atti di normazione secondaria, in particolare decreti ministeriali e interministeriali, che regolano gli aspetti di dettaglio della disciplina: molto lavoro è stato già compiuto e i competenti organismi tecnici ormai insediati sono attivamente impegnati per tale processo, anche al fine di recuperare i ritardi accumulatisi. Un passaggio essenziale sarà l'istituzione - ormai prossima - del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), la banca dati che dovrà riunire tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti. La mancanza di un quadro normativo compiutamente definito, soprattutto a causa dei ritardi nell'emanazione dei già citati atti di normazione secondaria, crea problemi sia agli enti istituzionali preposti alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali sia alle stesse parti sociali che quelle norme sono chiamate ad applicare. Occorre allora proseguire con impegno lungo questa strada, superando le resistenze e le difficoltà che ancora permangano, dovute soprattutto alla oggettiva complessità tecnica della materia e alla necessità di mettere d'accordo i tre diversi gruppi di soggetti ai quali la normativa stessa affida l'elaborazione delle disposizioni di dettaglio, ossia amministrazioni centrali, Regioni e parti sociali. La Commissione, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, intende proseguire il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Testo unico, confrontandosi direttamente con i vari soggetti coinvolti. Come è avvenuto finora, tale attività mira a valutare gli effetti concreti derivanti dalle nuove disposizioni, nonché ad individuare gli eventuali problemi applicativi e le possibili soluzioni. A tal fine, A tal fine, la Commissione si propone, in particolare, di continuare a svolgere sopralluoghi sul territorio, per acquisire informazioni dirette sulle modalità con le quali, nelle varie parti del Paese, si attuano concretamente le azioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale ambito, un'attenzione specifica sarà rivolta alle istituzioni regionali, alle quali la nuova normativa assegna un ruolo essenziale di coordinamento e di programmazione. L'attuazione della nuova disciplina presenta, infatti, ancora differenze e disomogeneità nelle varie parti d'Italia, che occorre cercare di superare. L'intento della Commissione è quindi, da un lato, quello di raccogliere utili elementi di conoscenza e di riflessione; dall'altro, quello di offrire un contributo di attenzione e di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti che operano in prima linea sul territorio. Questo tema si lega strettamente all'esigenza, già segnalata nella precedente relazione, di accrescere sempre più il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in ambito centrale che periferico. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha posto molta evidenza a tale aspetto, prevedendo tra l'altro appositi istituti per rafforzare la collaborazione fra i vari enti: in particolare, a livello nazionale il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e, a livello locale, i Comitati regionali di coordinamento (articolo 7). Come si è detto, l'insediamento e l'avvio delle attività di questi organismi ha dato risultati positivi, ma molto lavoro resta da fare. Fra i vari enti del settore, infatti, si registrano ancora casi di sovrapposizione e duplicazione di competenze, ad esempio in materia di ispezioni e controlli, che rallentano e indeboliscono i risultati dell'azione amministrativa. Già nella precedente relazione intermedia si è posto in evidenza come questo problema si leghi ad una esigenza più generale di riorganizzazione della pubblica amministrazione,

è rappresentato dal trasferimento in capo all'INAIL delle competenze prima attribuite all'IPSEMA e all'ISPESL, ma il dibattito politico e anche culturale su questi temi, certamente complessi, è quanto mai aperto e lungi dall'essere concluso. Nel frattempo, occorre rafforzare ulteriormente la collaborazione e la sinergia tra i diversi organismi statali e non statali per rendere sempre migliore, più univoco e più coerente il servizio offerto alla collettività (imprese, lavoratori e cittadini) in questo delicato settore. La Commissione continuerà ad offrire il proprio contributo a questo processo nel quadro delle proprie competenze istituzionali, favorendo la riflessione su questi temi e il dialogo tra le diverse amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, anche al fine di individuare soluzioni condivise per una eventuale riorganizzazione complessiva del settore, con particolare riguardo al tema della legislazione concorrente Stato-Regioni. Particolare attenzione deve poi essere dedicata ai controlli e alla repressione delle infrazioni, attraverso una applicazione equilibrata ma rigorosa delle sanzioni. Anche in questo caso l'azione sinergica degli organismi ispettivi, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, potrà dare risultati sempre migliori, specialmente, ma non solo, nel contrasto alle violazioni più gravi e pericolose. Le convenzioni recentemente stipulate dal Ministero del lavoro con l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza sono un importante esempio. La Commissione ritiene opportuno continuare con decisione lungo questo percorso, rafforzando la collaborazione e il coordinamento tra gli enti ispettivi nell'intento di accrescere l'efficacia dei controlli, razionalizzare gli interventi, assicurare modalità operative uniformi. La banca dati SINP potrà certamente dare un contributo essenziale in tale direzione, aiutando a programmare meglio gli interventi e la vigilanza su base territoriale ed eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.

Un altro aspetto cruciale per la promozione di una vera cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro è quello della formazione-informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, che deve essere impostata in un'ottica di prevenzione e con un approccio di tipo sistematico, multidisciplinare. L'indagine della Commissione, infatti, ha dimostrato come i risultati migliori in questo campo non derivino dalla mera trasmissione di nozioni tecniche, magari astratte, ma piuttosto da un approccio concreto volto a creare una consapevolezza, una *forma* *mentis* che accresca il livello di attenzione da parte dei singoli soggetti (lavoratori e datori di lavoro) e dell'intero contesto aziendale. Ciò implica un addestramento continuo, non limitato al momento dell'ingresso in un nuovo lavoro o settore produttivo e che dovrebbe anzi partire dalla scuola stessa, proprio per creare, fin dalla più giovane età, quella consapevolezza di cui si è appena detto. La Commissione, anche attraverso l'apposito gruppo di lavoro su formazione e prevenzione, intende proseguire nell'approfondimento di questi temi per focalizzare gli aspetti più critici e stimolare la ricerca di possibili soluzioni. In Italia, la formazione-informazione sui temi della sicurezza resta, infatti, problematica, in quanto non esiste ancora un numero sufficientemente elevato di corsi universitari sull'argomento e non tutte le Regioni hanno organizzato programmi adeguati. A tal fine, sono stati comunque stanziati appositi fondi per il triennio 2008-2010 nell'ambito delle azioni promozionali di cui all'articolo 11 del Testo unico, d'intesa con le Regioni e le parti sociali. Sebbene si tratti di risorse limitate, è tuttavia un segnale importante. Anche per quanto riguarda l'introduzione dei temi della sicurezza sul lavoro negli insegnamenti scolastici, l'apposita cabina di regia, costituita dal Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione ed INAIL, ha iniziato la propria attività solo recentemente. L'elaborazione delle linee guida e l'adozione dei necessari provvedimenti richiederà, quindi, ancora qualche tempo. La Commissione auspica che si prosegua con decisione lungo questa strada, rafforzando le iniziative già in corso e garantendo sufficienti risorse anche con il contributo delle organizzazioni sindacali edatoriali, da sempre molto attive su questo fronte. Essa ritiene altresì necessario che vengano definiti indirizzi aggiornati e omogenei sui contenuti e sulle modalità della formazione per il mondo scolastico e universitario, nonché per le iniziative di carattere privato, così da garantire insegnamenti adeguati da parte di esperti qualificati. Accanto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, la Commissione segue con attenzione anche le questioni legate alla prevenzione e al contrasto delle malattie professionali. È auspicabile che l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro possa aiutare l'emersione dei casi di malattia che, per varie ragioni, ancora sfuggono alla rilevazione - le cosiddette malattie perdute - e favorire così l'attività di prevenzione e di sorveglianza sanitaria. La Commissione auspica a tal fine il coinvolgimento sempre più ampio non solo dei medici competenti e specialistici, ma anche dei medici generici e di base, che hanno un controllo più frequente con i pazienti. Altrettanto auspicabile sono una presa di coscienza sempre maggiore da parte dei lavoratori ed uno snellimento delle procedure di riconoscimento e di indennizzo da parte dell'INAIL, soprattutto per le patologie non tabellate. Gli infortuni sul lavoro hanno spesso un carattere ripetitivo ed in molti casi potrebbero essere più facilmente prevenuti prendendo spunto dagli incidenti già accaduti. In questo senso è auspicabile che le varie banche dati già esistenti nonché il citato SINP possano essere utilizzate anche a tal fine e che le informazioni sugli incidenti occorsi nei vari settori possano, nel rispetto della *privacy* e degli eventuali segreti istruttori, essere messe a disposizione riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai fini della prevenzione. La Commissione ritiene opportuna l'introduzione di forme di incentivazione volte a premiare le imprese virtuose che investono nella sicurezza sul lavoro attraverso sgravi e agevolazioni fiscali e contributive. In questo ambito, essa auspica altresì la prosecuzione della concessione di incentivi per favorire la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione e causa di infortuni anche gravi. Appare soprattutto opportuno estendere le misure già previste per tali macchine e attrezzature anche alle cosiddette opere provvisionali dell'edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro), la cui efficienza ed adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli infortuni nel settore. Uno dei settori più critici per il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è certamente quello degli appalti, dove, malgrado l'esistenza di disposizioni assai avanzate, si riscontrano talora ribassi eccessivi nelle offerte sia per la realizzazione che per la progettazione dei lavori, con il rischio di comprimere i costi della sicurezza e di abbassare la stessa qualità delle prestazioni. Ciò accade soprattutto nel settore privato, dove non esistono regole cogenti in materia di appalti e molti operatori sono privi di adeguata qualificazione, nel caso delle piccole e piccolissime imprese appaltatrici, meno attente ai profili della sicurezza, e nelle catene più lunghe dei subappalti, dove i controlli sono più difficili e a volte si inserisce anche la criminalità organizzata. Nel settore pubblico, vi è poi la difficoltà di molte amministrazioni pubbliche appaltanti di valutare la congruità delle offerte e le giustificazioni delle eventuali anomalie addotte dalle imprese partecipanti alle gare, che spesso avviano lunghi e pesanti contenziosi. Per superare tale situazione, la Commissione ritiene essenziale, accanto ad un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni, un ripensamento della normativa vigente che, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e della libertà di impresa, fissi regole più certe e selettive, limitando il ricorso al massimo ribasso quale criterio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del subappalto. Occorre estendere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico, nonché, in quest'ultimo, rafforzare la capacità tecnica delle stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte

in collaborazione con le organizzazioni di categoria ed in stretto raccordo con i competenti Ministeri. In conclusione, signor Presidente, desidero ringraziare tutti i colleghi della Commissione, con i quali anche quest'anno abbiamo lavorato e collaborato. Desidero ringraziare coloro i quali coordinano i gruppi di lavoro, che nella nostra Commissione sono ben dieci, il

a competizioni che le diverse sensibilità politiche di ognuno di noi avrebbero potuto alimentare. Di questo ringrazio vivamente tutti i colleghi e spero che anche

Sono presenti in tribuna, in occasione della loro visita al Senato, gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giuseppe Montezemolo» di Roma. Rivolgiamo i nostri auguri per il nuovo anno e per l'attività di studio a loro e ai loro insegnanti.

sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro consente a quest'Aula di riflettere su uno dei temi più importanti e più drammatici che investono il nostro Paese: il continuo ripetersi di infortuni e decessi, anche se negli ultimi anni abbiamo potuto registrare un fenomeno decrescente sia degli infortuni sia dei decessi, dato che comunque va contestualizzato rispetto alla crisi economica, alla diminuzione dei posti di lavoro che ha investito il nostro Paese, che ha determinato una diminuzione sia delle ore lavorate sia del numero degli addetti. Per il 2009 sono stati censiti 790.000 infortuni e 1.050 decessi. Va poi notato che negli ultimi mesi, anche a causa di questa crisi economica e della disperazione che c'è in tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'attenzione sulle questioni della sicurezza viene a diminuire. Un dato questo che con tutta evidenza non è in alcun modo accettabile e che dovrebbe interrogarci tutti, politici, imprenditori, sindacati e pubblica opinione, su quanto ancora dovremo fare per debellare questa piaga: una tragedia quotidiana che rischia di offuscare i principi di civiltà

La Commissione d'inchiesta, in un clima collaborativo e costruttivo, ha svolto in questi mesi un proficuo lavoro di approfondimento, articolando la sua attività sia intervenendo direttamente nei luoghi dove dove si sono avuti incidenti più gravi, sia interloquendo coi soggetti e le amministrazioni addetti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno In particolare, dalla esperienza prodotta in questi mesi, ho maturato la convinzione che l'elaborazione di uno corpo normativo organico, se non accompagnata da risorse economiche adeguate per la ricerca, la prevenzione e la formazione e da personale qualificato addetto al monitoraggio e alla repressione degli abusi, non è sufficiente a reprimere il fenomeno. purtroppo, non posso non denunciare che su questo tema l'attuale Governo ha segnato dei passi indietro anche rispetto all'immediato passato. Come non possiamo non ricordare le modifiche apportate dall'attuale Governo al decreto legislativo n. 81 di risoluzione che, a parte il giudizio sull'operato del Governo, in gran parte converge col testo proposto dalla maggioranza, intendiamo chiedere garanzie al Governo nel merito: dell'emanazione del decreto attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto, come previsto dalla legge finanziaria 2008; del completamento, in tempi rapidi, dell'attuazione della riforma introdotta dal citato decreto legislativo n. 81, in particolare per l'avvio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in modo da offrire a tutti i soggetti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (imprese, lavoratori, enti istituzionali) un quadro normativo completo ed un'applicazione uniforme delle disposizioni; del reperimento delle risorse; dell'assunzione di personale qualificato per rendere più incisivi i controlli e la repressione delle infrazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro

di promuovere norme in positivo, tese a premiare le imprese virtuose che investono nella sicurezza sul lavoro; di promuovere, come più volte richiesto unitariamente anche con atti di indirizzo della stessa Commissione, incentivi economici per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine ed attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette opere provvisionali dell'edilizia, (impalcature, ponteggi, piani di lavoro), la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli infortuni In particolare, però, vorrei soffermarmi su tre temi che sono stati spesso affrontati dalla Commissione, anche nel confronto diretto con il Ministro del lavoro. il tema degli appalti e dei subappalti nel settore pubblico, e anche privato, che rischiano, con il principio del massimo ribasso, di scaricare i costi e i danni della sicurezza sui lavoratori e che penalizzano le imprese sane ponendole fuori dal mercato degli appalti. Si tratta di un tema particolarmente serio, che incide direttamente sulla prassi per la sicurezza e che spesso rende particolarmente difficile individuare le responsabilità. Vi è poi il tema del coordinamento e dell'unificazione delle normative antinfortunistiche sull'intero territorio nazionale. La sicurezza sul lavoro, a mio avviso, non può che essere assicurata a livello nazionale: le competenze delle Regioni sono altre, vanno rispettate e anche aumentate, ma in questo caso non possono esistere più legislazioni. Credo che le stesse Regioni siano sensibili al tema, perché hanno compreso che un conto è la legislazione, altro conto sono i poteri loro assegnati. modo, dovremmo arrivare a definire sedi di coordinamento tra vigili del fuoco, ASL, ispettori del lavoro, NAS e quant'altri. Infine - anche a partire dall'esperienza maturata nel corso dell'ultima missione

attraverso una più efficace formazione ed un rafforzamento dei controlli e delle correlative sanzioni a carico delle imprese inadempienti e la predisposizione di un piano di bonifiche soprattutto di siti abusivi da dove emergono sversamenti di materiali tossici, ed in particolare di rifiuti contenenti amianto; a favorire l'adeguamento colgo l'occasione di questo dibattito in Aula per richiamare tutti alla centralità di questo tema, perché esso non venga relegato, come spesso accade, ai cosiddetti esperti del settore.

È un tema che bisogna ricordare sempre, per prevenire e intervenire. Tengo inoltre a sottolineare il clima di collaborazione che in questi mesi ha contraddistinto il lavoro della Commissione, l'equilibrio dimostrato dal Presidente, e anche la particolare professionalità

spero si possa giungere, al di là di un diverso giudizio sul Governo, che noi ovviamente abbiamo ribadito e ribadiamo, all'approvazione unitaria di un dispositivo che tenga conto di questo lavoro e indichi la prospettiva da seguire nel prossimo anno.

ben illustrata dal senatore Nerozzi, in Italia ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti sul lavoro. Anche nel 2009, voglio anch'io sottolinearlo, nonostante la grave crisi economica che ha comportato una significativa riduzione delle ore lavorate, ci sono stati 790.000 infortuni, di cui 1.050 mortali. Una piaga sociale inaccettabile per un Paese civile come l'Italia; un Paese, il nostro, dove i diritti in materia di sicurezza sul lavoro sovente sono In particolare, ciò che maggiormente colpisce sono le cause principali di questi numerosi infortuni: cause spesso ripetitive, come le cadute dall'alto nel settore dell'edilizia, l'asfissia dei lavoratori adibiti alla manutenzione delle cisterne, oppure, come accaduto due mesi fa in un'azienda per il trattamento dei rifiuti industriali in provincia di Milano dove c'è stato un incidente spaventoso che ha provocato la morte di due lavoratori e il ferimento di altri cinque, di cui due versano ancora

Tutti incidenti, come dicevo, dal carattere ripetitivo, assolutamente evitabili attivando misure di sicurezza elementari, come, ad esempio, le le protezioni per impedire le cadute dall'alto, la dotazione di autorespiratori per chi entra in cisterne chiuse da bonificare e soprattutto l'informazione e la formazione dei lavoratori in ordine ai rischi caratterizzano l'attività lavorativa e alle misure da adottare per la loro prevenzione. A quest'ultimo riguardo mi sembra opportuno segnalare che uno dei principali problemi che ostacolano una corretta informazione comprensione della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri. Infatti, come ha recentemente sottolineato la procura di Milano, «il lavoratore che non comprende l'italiano non può essere non si può considerare informato. È quindi del tutto evidente che nell'attività di informazione e di formazione di questi lavoratori deve essere assolutamente accertata la conoscenza della nostra lingua. Insieme al problema degli infortuni, come sottolineava il relatore Tofani, c'è anche quello delle malattie professionali, un fenomeno ed è proprio per questa ragione che la proposta di risoluzione che abbiamo presentato sottolinea la necessità di assumere iniziative adeguate per favorire l'emersione delle malattie professionali ancora non rilevate (le cosiddette malattie perdute). A questo proposito è davvero auspicabile che l'istituzione del Sistema informativo nazionale

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del Senato sulle difficoltà che incontrano i lavoratori, non solo rispetto al riconoscimento ed equo risarcimento dei danni da lavoro, ma anche nel reintegro al lavoro allorché abbiano subito menomazioni, sia in conseguenza di malattie da lavoro che di infortuni. In questo caso

dei lavoratori dopo una malattia o un infortunio sul lavoro, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 gennaio 2008. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

altrimenti si creano problemi e difficoltà agli enti preposti alle azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

attivano concretamente per mettere in campo le azioni di tutela della salute e della sicurezza.

presso gli stabilimenti ThyssenKrupp di Terni, la DSM di Capua, l'EURECO - caso prima richiamato - di Paderno Dugnano, il porto di Genova, i cantieri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, l'ENEL di Civitavecchia,

per analizzare e approfondire il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ma, soprattutto, per indicare le misure preventive. Ovviamente, questo importante impegno

le risoluzioni presentate sono indicate con chiarezza quali sono le azioni che il Governo deve mettere in campo con la massima tempestività. Ci aspettiamo quindi, signor Presidente, signor ministro Sacconi, impegni concreti e soprattutto risorse adeguate affinché le amministrazioni centrali e territoriali siano messe nelle condizioni di superare le criticità del sistema di prevenzione e di repressione che finora hanno impedito di combattere con efficacia questo grave fenomeno sociale.

considerato che in Italia ogni anno continua a registrarsi un alto numero di infortuni e di morti sul lavoro, inaccettabile in un Paese sviluppato, pari a 874.940 casi di infortunio (di cui 1.120 mortali) nel 2008 e 790.000 casi di infortunio (di cui 1.050 mortali) nel 2009; Tale dato, che ad una lettura superficiale potrebbe apparire come segnale di un *trend* decrescente del fenomeno (che peraltro da dati non ufficiali del 2010 sembrerebbe di nuovo in crescita), in realtà non tiene conto di fattori quali la diminuzione delle ore lavorate in conseguenza della contrazione della produzione industriale causata dalla crisi economica e il fenomeno delle mancate denunce degli infortuni da parte di categorie deboli di lavoratori quali immigrati e precari. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, il cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, l'Italia era stata finalmente dotata di una legislazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite la razionalizzazione e l'innovazione dell'assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico completo ed esaustivo nella definizione di istituti, soggetti e funzioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro e rigoroso nelle eventuali sanzioni da comminare. Tale disciplina risultava sicuramente esaustiva ed in linea con gli standard giuridici comunitari ed internazionali, come la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso di una missione conoscitiva compiuta nell'ottobre 2008 in Francia, Germania e Regno Unito. Con il decreto legislativo n. 106 del 2009 ed una lunga serie di altre disposizioni contenute in vari provvedimenti, il Governo è intervenuto sul testo unico del 2008, in particolare per quanto concerne le norme in tema di controlli, smantellandone di fatto il rigoroso impianto sanzionatorio. Al fine di garantire quel minimo di efficacia che la disciplina attuale può assicurare, è necessaria, almeno, una sua rapida e puntuale attuazione accompagnata da controlli rigorosi e da un costante monitoraggio. Come rilevato dalla Commissione, sono dunque ancora molte le criticità del sistema della prevenzione e della repressione del fenomeno infortunistico che rendono necessari forti interventi normativi correttivi e migliorativi. Per questa ragione, la proposta di risoluzione del Gruppo dell'Italia dei Valori impegna il Governo: ad assicurare il completamento, in tempi rapidi, dell'attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, anche alla luce delle successive modificazioni e integrazioni, procedendo all'adozione dei vari atti di normazione secondaria tra i quali, in particolare, quelli necessari per l'avvio del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il cosiddetto SINP); ad accrescere il coordinamento e le sinergie fra tutti gli enti istituzionali preposti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in ambito centrale che periferico, secondo quanto espressamente previsto dal decreto legislativo n. 81 ad adoperarsi, attraverso la destinazione di congrui stanziamenti di risorse economiche ed umane, affinché i soggetti preposti al monitoraggio circa la corretta applicazione della normativa e alla segnalazione e repressione di eventuali violazioni della normativa stessa siano posti nella condizione di espletare pienamente le proprie funzioni, rendendo più incisivi i controlli e la repressione (con particolare riguardo ai fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, nonché dello sfruttamento del lavoro minorile), attraverso un'applicazione rigorosa delle sanzioni e il coordinamento di tutti gli organi ispettivi, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, nell'intento di razionalizzare gli interventi ed assicurare procedure e strumenti di verifica uniformi; a favorire un'incisiva azione di monitoraggio dei singoli settori lavorativi, anche attraverso l'istituzione di appositi centri regionali, al fine di individuare per ciascuno di essi gli strumenti, anche economico-finanziari, più idonei a favorire il perseguimento della sicurezza sul lavoro; a favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in modo particolare attraverso l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di moduli didattici relativi ai temi della salute e della sicurezza, e soprattutto favorendo la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro con particolare attenzione al settore delle piccole e medie imprese; a destinare risorse finalizzate alla sicurezza degli edifici pubblici, in particolar modo di quelli scolastici, attraverso la sistemazione delle strutture pericolanti e la rimozione di sostanze o fibre pericolose per la salute delle persone, come l'amianto; ad assumere le iniziative necessarie per favorire l'emersione delle malattie professionali ancora non rilevate (le cosiddette malattie perdute) e le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria, anche attraverso il coinvolgimento dei medici generici e di base; a promuovere iniziative volte all'individuazione e alla prevenzione delle cause degli incidenti mancati per casi fortuiti; a rendere disponibile, nel rispetto della *privacy* e degli eventuali segreti istruttori, le informazioni sugli incidenti ripetitivi e più frequenti occorsi nei vari settori, con riguardo ai dati tecnici e a tutti gli aspetti utili ai fini di una migliore prevenzione; ad introdurre forme di incentivazione volte a premiare le imprese virtuose che investono nella sicurezza sul lavoro attraverso sgravi e agevolazioni fiscali e contributive, nonché a proseguire la concessione di incentivi per la rottamazione e la messa in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole, forestali ed edili, spesso obsolete ovvero prive di adeguati dispositivi di protezione, estendendole anche alle cosiddette "opere provvisionali" dell'edilizia (impalcature, ponteggi, piani di lavoro), la cui efficienza e adeguatezza sono essenziali per la prevenzione degli infortuni del settore; ad assumere adeguate iniziative legislative e amministrative, nel rispetto delle disposizioni comunitarie

fissando regole più certe e selettive, non perseguendo il ricorso al massimo ribasso quale criterio di valutazione delle offerte, accrescendo la qualificazione delle imprese e contenendo la pratica del subappalto. al fine di contrastare il deleterio fenomeno per cui l'abbattimento dei costi volto a garantire offerte più competitive si traduce spesso, da parte delle imprese più sleali e spregiudicate, in una riduzione delle spese per la sicurezza, e quindi, in un pericoloso abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori, oltre che in un peggioramento della qualità stessa dell'opera L'obiettivo è quello di estendere, per quanto possibile, anche al settore privato le garanzie e i controlli vigenti nel settore pubblico a regolamentare l'accesso all'attività di imprenditore edile (e, in particolare, la relativa iscrizione alla Camera di commercio) in modo da garantire adeguati e comprovati requisiti di professionalità, organizzazione ed esperienza per lo svolgimento dell'attività stessa; stessa; a fare in modo che, nei luoghi colpiti da calamità naturali, i macchinari e le attrezzature recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo siano sottoposti gratuitamente alle necessarie verifiche tecniche da parte dei competenti organismi di controllo, anche e soprattutto al fine di assicurare la loro idoneità

Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, l'impegno di questa Commissione volge ad oggi ad un nodo fondamentale. Siamo infatti in procinto di mettere a punto la relazione finale che raccoglierà tutti i dati raccolti sia nelle audizioni svolte in questa sede, che attivamente nelle missioni nazionali e internazionali. Ringrazio il presidente Tofani e tutti i colleghi per la collaborazione durante questo percorso fortemente impregnato di serietà e passione, ma soprattutto per la grande volontà di migliorare il nostro Paese sul piano del lavoro e della sicurezza sul lavoro. Questo è sempre stato l'obiettivo della Commissione cui ho l'onore di prendere parte. abbiamo cercato di approfondire alcuni aspetti per fornire al Parlamento e al Governo un migliore quadro conoscitivo della situazione del nostro Paese sul fronte lavoro, tutela del lavoro e sicurezza dei lavoratori. Tale Commissione ha svolto 57 audizioni, 15 missioni conoscitive di cui una all'estero e 14 in Italia; al suo interno sono stati costituiti gruppi di lavoro tematici al fine di approfondire specifici argomenti o problemi settoriali. Nella fattispecie il gruppo di lavoro cui sono chiamata a partecipare si è concentrato ed ha avuto modo di approfondire il tema dello sfruttamento minorile e quello del lavoro sommerso con risultati importanti. L'esito delle ricerche, delle audizioni e delle missioni ha mostrato una brutale realtà. In primo luogo, ha evidenziato la fortissima presenza di lavoro minorile e di abbandono della scuola dell'obbligo con percentuali elevate soprattutto nel Sud Italia. Ancora più preoccupanti sono l'incongruenza e l'imprecisione dei dati inviatici dagli enti preposti a tali accertamenti. Allo scopo di visionare questa situazione sono state messe sotto osservazione quattro Regioni il cui stato è considerato particolarmente critico: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. In secondo luogo, e non meno importante, ha evidenziato la presenza di lavoro sommerso e quindi la scontata relazione tra questa tipologia di rapporto lavorativo assolutamente non tutelata e la frequenza di infortuni sul lavoro. Molto è stato fatto grazie alla continua osservazione del fenomeno da parte di questa Commissione, alle continue audizioni degli enti preposti, alla creazione di reti e di scambi di informazione tra tali enti e alle missioni e ispezioni *in loco*, ma molto resta ancora da fare sia a livello legislativo sia dal punto di vista operativo per garantire al lavoratore il massimo della tutela e ai giovani il diritto allo studio così come garantito dai nostri principi fondamentali. Abbiamo apprezzato i fondi messi a disposizione dall'istituto INAIL, finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. La somma stanziata ammonta a 60 milioni di euro: spero sia un primo passo per le nostre imprese, che stanno attraversando un periodo molto particolare. particolare. Auspico, pertanto, una sempre maggiore attenzione al problema in analisi e che gli si garantisca e gli si continui a garantire un giusto spazio nel lavoro della nostra Commissione. *(Applausi

dal senatore Roilo. Ricordo come uno dei punti in questione riguardi la tutela della salute dei lavoratori, nello specifico la sorveglianza sanitaria che dovrebbe essere garantita in forma gratuita anche ai lavoratori che hanno cambiato lavoro o sono stati collocati in pensione dopo essere stati esposti all'amianto o ad altre sostanze cancerogene, genotossiche o teratogene. Altra questione è quella che concerne i controlli e la repressione delle infrazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al fenomeno del lavoro sommerso e allo sfruttamento del lavoro minorile. Come ben segnalato dalla Commissione, la necessaria attività di coordinamento tra tutti gli organi ispettivi. Mi preme sottolineare come, durante l'audizione del procuratore generale di Firenze davanti alla Commissione, il 24 febbraio 2010, sia stata rilevata la diffusa impreparazione della magistratura, requirente e giudicante, per quanto concerne la specializzazione per la trattazione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È stata inoltre segnalata la scarsa diffusione, salvo lodevoli eccezioni, di iniziative di coordinamento tra procure e organi di vigilanza delle ASL. Anche per conoscenza diretta, rilevo inoltre come vi sia il misconoscimento di una norma approvata dal Parlamento quando si discusse del disegno di legge in materia di sicurezza in senso lato. Avevamo infatti introdotto criteri di priorità per la trattazione di indagini e processi relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, ma di tale disposizione parlamentare pare che la magistratura, per la gran parte, si disinteressi. Anche questo dato relativo a criteri di priorità va assolutamente segnalato.

più ampia possibile, la pratica del subappalto, in particolare non perseguendo il ricorso al massimo ribasso come criterio di valutazione delle offerte, perché è per tutti comprensibile

*(PdL)*. Signor Presidente, per prima cosa vorrei ringraziare personalmente il presidente Tofani, che ha coordinato i lavori della nostra Commissione con equilibrio e moderazione, dando ascolto alle voci di tutti e creando un clima di lavoro positivo da cui tutti noi abbiamo tratto giovamento. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro si è occupata sin dall'inizio della XVI legislatura di incidenti in ambito domestico, istituendo un apposito gruppo di lavoro, acquisendo i dati necessari alla comprensione della reale situazione e ascoltando i pareri e le analisi di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella cura dell'infortunio in casa. La legge n. 433 del 1999 ha equiparato, in linea di principio, il lavoro domestico a qualsiasi altra attività lavorativa, riconoscendo dunque pari dignità al lavoro di oltre cinque milioni di casalinghe. La legge ha poi istituito un sistema di raccolta dati presso l'Istituto superiore di sanità, stabilendo l'obbligo di assicurazione per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente da lavoro svolto in ambito domestico, dando all'INAIL, ai Ministeri competenti e alle associazioni di categoria la responsabilità di gestire un fondo autonomo speciale che ha il compito di raccogliere i premi e pagare le rendite. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge è stato necessario tracciare un bilancio: la legge n. 433 del 1999 non ha ridotto gli infortuni in ambito domestico e l'assicurazione obbligatoria vive una situazione di stallo preoccupante. Risultati positivi sono riscontrabili solo nella raccolta dati e nell'analisi del fenomeno. In altre parole, adesso abbiamo un quadro più chiaro sugli infortuni domestici. Inoltre, i progressi tecnologici e le scoperte in campo scientifico hanno reso più sicure le cucine (dove avviene il 58 per cento degli incidenti che coinvolgono le donne), gli impianti di riscaldamento e gli elettrodomestici, ma non hanno ridimensionato significativamente il numero di infortuni. Il numero dei morti a seguito di incidente in ambito domestico è ancora molto elevato. Il dato non è uniforme né oggettivo in quanto ogni istituto di ricerca utilizza metodologie differenti di classificazione: secondo l'Istituto superiore di sanità i decessi sarebbero 5.500, secondo l'Istituto nazionale lavoro (ISPESL) 7.500. Gli infortuni, di ogni entità, sono ben oltre tre milioni l'anno. Le principali cause di incidente sono per la maggior parte le cadute seguite da tagli e punture, urti e schiacciamenti, ustioni, soffocamenti e avvelenamenti. L'80 per cento dei casi di soffocamento riguarda le donne, i casi di folgorazione riguardano donne per il 70 per cento, e i casi di ustione riguardano donne per il 60 per cento. Esiste dunque una condizione di rischio assimilabile al rischio professionale presente in un'industria o in una fabbrica. L'esposizione a sostanze tossiche, così come l'utilizzo di apparecchi domestici, è un problema serio che espone la casalinga ad un rischio di breve termine legato soprattutto all'uso di sostanze caustiche, ma anche ad un rischio a lungo termine ancora poco studiato. Il numero di decessi e infortuni in casa è dunque estremamente preoccupante nonostante il livello di allarme sociale sia molto basso. La percezione di casa come luogo sicuro aumenta inoltre il rischio di infortunio se si considera che le principali cause di incidente sono la distrazione e l'inappropriatezza dei comportamenti più che il mal funzionamento degli elettrodomestici o degli impianti a gas. È chiaro che tutto questo non è accettabile e che le cose devono cambiare. Dai dati presentati emerge la necessità di concentrare gli sforzi del legislatore sulla prevenzione. Per le donne in età lavorativa è stata studiata la possibilità di inserire nei corsi pre-parto alcuni incontri di formazione sugli infortuni domestici, mentre per la fascia di età più elevata gli strumenti predisposti appaiono scarsamente efficaci. In particolare, opuscoli informativi (spesso complicati) o pubblicazioni scientifiche *on line*, pur se facilmente reperibili, vengono in realtà consultate solo dagli addetti ai lavori. Per questa fascia di età bisogna passare attraverso i centri anziani presenti sul territorio e soprattutto attraverso la televisione nazionale e locale che è in grado di veicolare il messaggio anche presso le persone che vivono in condizione di emarginazione e solitudine. Le risorse per incrementare l'attività di prevenzione non mancano, ma l'erogazione di rendite si è praticamente bloccata e le casalinghe continuano a pagare i premi assicurativi senza di fatto ricevere né il risarcimento in caso di infortunio né un'adeguata attività di prevenzione. Dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2009 sono state presentate oltre 10.000 domande di rendite, delle quali solo 581, sono state accettate: poco più del 4 L'assicurazione obbligatoria, invece, riguarda le persone in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono attività in ambito domestico per la cura del nucleo familiare e dell'abitazione e che non siano impegnate in altra attività lavorativa. Secondo l'INAIL, sono 5 milioni e 200.000 le persone che rientrano in questa categoria, ma al 31 dicembre 2008 risultavano iscritti solo poco più di 2 milioni di soggetti con differenze su base regionale. Essendo il premio già particolarmente basso (appena 12 euro e 91 centesimi), i motivi per i quali la metà delle casalinghe non si assicura sono solo la scarsa conoscenza della norma e la scarsa fiducia nei confronti dell'INAIL che rigetta quasi il 90 per cento delle richieste di risarcimento. A seguito delle audizioni dei rappresentanti di INAIL, ISPESL e ISS in Commissione infortuni, cento delle domande viene rigettato in quanto l'invalidità cagionata da incidente domestico è al di sotto della soglia fissata per legge. L'abbassamento del grado minimo di indennizzabilità dal 33 cento disposto dalla finanziaria del 2007 non è stato sufficiente ad aumentare considerevolmente il numero delle rendite pagate. Quella degli infortuni sul lavoro è, in generale, una delle piaghe che più colpisce il nostro Paese e che viene spesso trascurata anche dai mezzi di informazione, i quali preferiscono dare spazio a notizie più sensazionalistiche che catturano di più l'immagine dei lettori e dei telespettatori, non cogliendo il dramma di chi - sia esso imprenditore o lavoratore dipendente - esce di mattina per andare a svolgere la sua attività senza poi rientrare a casa la sera. Il lavoro di questa Commissione, in tutte le sue componenti, maggioranza e opposizione, è stato assiduo e proficuo durante questi primi due anni e mezzo. Lo dimostrano la relazione, votata all'unanimità dalla Commissione stessa, e l'atteggiamento positivo di tutti i membri con i quali ho avuto il piacere di collaborare. Spesso, per cambiare le cose, basterebbe poco. Basterebbe che gli operai iniziassero a utilizzare il caschetto con maggiore frequenza - come le cinture di sicurezza per le macchine - nei cantieri edili. Ma sono convinta che, siccome gli infortuni stanno già calando (sebbene in questo caso una sola vittima è sempre di troppo), con l'impegno di tutti noi in Parlamento, delle parti sociali e delle altre istituzioni, tra cui è doveroso ricordare il Presidente della Repubblica che da tempo cerca - giustamente - di catturare l'attenzione della nostra popolazione su questo tema, potremo sconfiggere questo problema, per il quale solo in questi anni ci si sta battendo con forza e determinazione. Signor Presidente, il problema delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro e soprattutto quello delle cosiddette morti bianche rimane un connotato negativo delle società avanzate *post* industriali ancora oggi, all'inizio del terzo millennio. In Italia, nell'ultimo decennio, il fenomeno ha registrato una sensibile riduzione, ma il numero degli infortuni e quello di lavoratori che perdono la vita in circostanze collegate allo svolgimento del proprio lavoro rimane pur sempre molto elevato. Secondo i dati diffusi nelle statistiche ufficiali relative al 2009, nel nostro Paese si sono avuti quasi 800.000 infortuni sul lavoro e, di questi, oltre 1.000 sono risultati mortali per le persone coinvolte. Rispetto al 2008 la riduzione è stata di quasi il 10 per cento per il totale degli infortuni e di oltre il 6 per cento per il numero di morti. Si tratta di una riduzione importante, perché conferma un *trend* in diminuzione che abbraccia l'intero decennio. Infatti, nel periodo che va dal 2002 al 2009, il calo complessivo è stato del 20 per cento degli infortuni totali e di quasi il 30 per le morti sul lavoro. Ma questi dati, certamente positivi e incoraggianti, non debbono indurci certo ad abbassare la guardia. Basta infatti esaminarli più in dettaglio per scoprire che il fenomeno delle morti bianche è ancora pieno di insidie e di trappole. Tanto per fare un esempio, il calo degli infortuni totali ha riguardato in larga parte gli uomini e molto meno le donne, le quali quindi rimangono evidentemente molto esposte ai rischi nello svolgimento delle loro attività quotidiane di lavoro. Nel settore edilizio, così come nell'agricoltura (settore dove la presenza del lavoro sommerso e nero è prevalente), la diminuzione dei morti sul lavoro è stata molto contenuta, poco sopra l'1 per cento, a fronte delle ampie riduzioni registrate negli altri settori. Infine, anche l'analisi del dato a livello territoriale conferma la storica sperequazione tra Centro-Nord, dove il numero di infortuni si riduce di più, e Mezzogiorno, dove il *trend* di riduzione è molto meno marcato. In linea generale, poi, non dobbiamo dimenticare che la riduzione così marcata degli incidenti sul lavoro registrata negli ultimi due anni è anche la conseguenza della crisi economica, che ha fatto ridurre la produzione. Non a caso la riduzione maggiore degli infortuni è stata registrata proprio nell'industria manifatturiera, più colpita dalla crisi rispetto agli altri settori. E questo aspetto ridimensiona certamente i risultati pur molto importanti delle politiche messe in campo, i quali sono sicuramente incoraggianti ma che lasciano poco spazio a facili trionfalismi. In questo contesto la Commissione parlamentare d'inchiesta si è posta l'obiettivo di indagare non solo sugli aspetti più comuni della problematica, cioè la dimensione del fenomeno, le sue cause, i costi impliciti per la finanza pubblica e gli eventuali nuovi provvedimenti legislativi da adottare, ma anche quello di indagare su aspetti forse meno blasonati, ma importantissimi, tanto per comprendere veramente a fondo il fenomeno quanto per individuare poi le azioni più opportune da mettere in campo per fronteggiarlo nel modo più efficace possibile. Tra questi aspetti giova ricordare in particolare: il grado di coinvolgimento negli incidenti dei minori, dei lavoratori precari e dei lavoratori di provenienza extracomunitaria; quanto rileva la presenza delle infiltrazioni della criminalità nelle imprese coinvolte; l'idoneità dei controlli messi in campo per ottemperare all'applicazione della normativa in vigore;

e sull'acquisizione di documenti, ma anche svolgendo sopralluoghi nelle località dove sono avvenuti gli incidenti più gravi e drammatici, per intervistare coloro che hanno visto e che hanno vissuto i fatti perché direttamente interessati, come datori di lavoro e lavoratori. Dalle visite *in loco* si è potuto acquisire un insieme di informazioni e di dettagli per mezzo dei quali si è costruito un quadro della situazione molto più completo di quello emergente dai soli dati statistici di sintesi: quadro che si è rivelato un complemento di fondamentale importanza ai risultati dello studio del sistema normativo e amministrativo che in Italia presidia la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quest'ultimo studio è stato, invece, realizzato principalmente per mezzo delle audizioni dei soggetti istituzionali e dell'acquisizione di documenti. Proprio grazie ai sopralluoghi si è potuto prendere atto di come le circostanze nelle quali maturano gli incidenti più gravi siano il frutto della complessità delle situazioni e delle operazioni svolte. Tale complessità deriva da un lato dall'essenza stessa della moderna produzione industriale, ma dall'altro anche dai molteplici rapporti contrattuali che si instaurano tra il committente e chi svolge effettivamente il lavoro. I predetti rapporti contrattuali, a volte non molto trasparenti, determinano una complessa e a volte minuziosa ripartizione dei singoli compiti all'interno della rete della produzione, alla quale, invece, non sempre fa seguito una altrettanto attenta e chiara attribuzione delle responsabilità. Questo tema specifico è stato oggetto di un approfondimento particolare della Commissione per quanto riguarda la correlazione degli incidenti con le pratiche di appalto e subappalto. Questa specifica analisi ha confermato il fatto che, specialmente negli appalti di grandi dimensioni, l'impresa appaltatrice principale si serve di una catena di imprese subappaltatrici che si trasferiscono tra di loro le singole parti dell'opera da realizzare. Nei vari passaggi però (e questo è in gran parte legato alle procedure di selezione delle imprese che sono basate sulle aste al massimo ribasso) gli aspetti di cura della sicurezza sono quelli sui quali si presta meno attenzione, vuoi perché l'appaltante tende a scaricare l'onere dei controlli sul subappaltatore, vuoi perché sono proprio i costi della sicurezza, purtroppo, quelli sui quali si tende a risparmiare di più. Gli effetti nefasti di queste pratiche sono spesso sulla cronaca e il lavoro della Commissione li mette oggi davanti agli occhi di tutti i componenti di quest'Assemblea. Per contrastare efficacemente il fenomeno degli infortuni sul lavoro occorre affiancare alla puntuale e corretta applicazione della normativa un'azione di costante monitoraggio delle situazioni più a rischio. Una corretta applicazione della normativa richiede il completamento in tempi rapidi della riforma introdotta con il decreto legislativo n. e cioè in via prioritaria l'emanazione della normativa secondaria di attuazione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale per la prevenzione. Per assicurare una azione di costante ed efficace monitoraggio bisogna coinvolgere nel modo più opportuno i soggetti responsabili del sistema dei controlli sul territorio, non solo le prefetture e le forze dell'ordine, ma anche i medici di medicina generale, da coinvolgere, questi ultimi soprattutto, nella parte che riguarda le malattie professionali, al fine di creare la consapevolezza in chi lavora e vi è esposto e quindi assicurare una migliore prevenzione. Già in sede di approvazione della prima relazione intermedia della Commissione abbiamo avanzato alcune specifiche proposte in tema di attività di vigilanza e prevenzione,

l'esigenza di rafforzare in maniera sempre più incisiva il coordinamento e la collaborazione fra tutti gli enti istituzionali che si occupano, a vario titolo, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia a livello centrale che locale, secondo quanto espressamente previsto dal Testo unico. In taluni casi, infatti, in questo campo si rileva ancora una sovrapposizione e duplicazione di competenze, ad esempio nella fase ispettiva e di controllo, che certamente non aiuta l'efficacia e la speditezza dell'azione amministrativa. Si tratta, per la verità, di un problema annoso, che si ricollega, da un lato, a quello più generale di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assistenziali

Si potrebbe lavorare immediatamente alla elaborazione di procedure standardizzate per la redazione di linee guida finalizzate alla stesura del verbale unico ispettivo, utilizzabile dagli organi preposti al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente. Oggi, lo ricordo, gli organi ispettivi di vigilanza dispongono di modelli in bianco, da compilare in maniera discrezionale nell'ambito delle ispezioni nei luoghi di lavoro. La pianificazione dei modelli standardizzati per la stesura dei verbali ispettivi, adottabili dagli organi competenti, garantirebbe anche una migliore efficacia nell'ambito del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 8 del Testo unico.

Un altro aspetto fondamentale è la formazione, su cui abbiamo lavorato molto. La Commissione ha ribadito la propria profonda convinzione della necessità di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza all'interno della scuola, come passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. Oltre che all'encomiabile processo avviato dal Ministero dell'istruzione e previsto dal citato articolo 11 n. 81, ritengo che il Ministero dell'istruzione debba avviare un piano di formazione integrato, in grado di dare assistenza e supporto ai dirigenti scolastici in maniera esaustiva per quanto concerne l'assolvimento dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza. Mi riferisco ai corsi di formazione per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, per i dirigenti, per i preposti, per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e per gli addetti ai servizi antincendio e primo soccorso.

proposito, riteniamo che il programma di azioni da intraprendere debba prevedere i seguenti capisaldi: la programmazione immediata degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; piani organici per la manutenzione degli edifici scolastici; l'attivazione urgente della normativa inerente il fascicolo del fabbricato per gli edifici scolastici (ricordo che oltre l'80 per cento delle scuole italiane non sono a norma per quel che riguarda la sicurezza nelle sue varie accezioni); verifica della ricettività degli edifici scolastici e razionalizzazione dei processi funzionali e degli spazi disponibili; la promozione di incisive iniziative di raccordo, coordinamento e cooperazione tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali, finalizzate agli scambi di informazioni, alla programmazione e gestione degli interventi di cui ai punti precedenti. Ricordo solo che il fascicolo del fabbricato è un documento che stabilisce la revisione dell'edificio per quanto concerne la sicurezza statica delle strutture e degli impianti, che dovrebbe essere adottato per tutti gli edifici del territorio nazionale. Chiediamo che venga redatto almeno per gli edifici scolastici ed i servizi Questa proposta, se adottata, rappresenterebbe un segnale forte da parte del Governo; oltre ad essere una risposta etica al fenomeno della insicurezza nelle scuole,

intendo anch'io ringraziare innanzitutto il presidente Tofani e i componenti tutti della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro sul lavoro per il lavoro comune svolto: un lavoro rilevante, importante, produttivo e sostanziale. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro ed alle morti bianche evidenziano, per il 2009, 790.000 incidenti sul lavoro, a fronte degli 875.000 del 2008; I dati, rapportati a quelli degli anni precedenti, sembrano confermare che il fenomeno degli incidenti e delle morti sui luoghi di lavoro sia in costante anche se lenta diminuzione. È anche vero che molti contestano questo apparente andamento "positivo", poiché a loro dire il dato relativo alla diminuzione di incidenti e di morti sui luoghi di lavoro va letto sia in relazione alle diminuite ore lavorate, sia in relazione ad una precarietà e ad una disoccupazione crescente che porterebbero di fatto a mancate denunce di infortuni. Ciò che appare comunque certo ed oggettivamente incontestabile è che 790.000 incidenti sul lavoro e 1.050 morti sono assolutamente e tragicamente troppi. E questo ancor più quando si considera il dramma che vi è dietro ognuno di quegli incidenti, il dramma che c'è dietro ognuno di quelle morti sul lavoro. Un incidente ogni 15 lavoratori, un morto sul lavoro ogni 8.100 addetti: queste, le cifre del fenomeno secondo l'Eurispes. Sono cifre superiori o paragonabili a quelli delle morti nelle guerre Dall'aprile 2003 all'aprile 2007, nella seconda guerra del Golfo, morirono 3.520 militari della coalizione, mentre dal 2003 al 2006 i morti sul lavoro sono stati ben 5.252. Cifre da guerra, appunto! Ma l'Italia non ha combattuto alcuna guerra. Il dramma però c'è, ed è continuo nella sua tragicità. È il dramma del lavoratore, delle famiglie che perdono un padre, un marito, un figlio: famiglie che al dolore per la perdita della persona cara o per la sua infermità debbono in molti casi sommare un calvario fatto di battaglie legali, burocrazie e difficoltà economiche. Sono ancora troppi gli infortuni e le morti sul lavoro. Sono troppi i circa 25.000 lavoratori che nell'anno appena trascorso sono rimasti invalidi per incidenti sui posti di lavoro; troppi in relazione al costo sociale che accompagna tale fenomeno. Costo sociale a carico di tutti, nessuno escluso; le assenze derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali i conseguenti costi economici correlati incidono infatti sia sull'economia, sia sulla competitività delle imprese. Costo sociale che, vorrei ricordare, è stato stimato in 45 miliardi di euro (anno 2005, ultimo dato INAIL disponibile), pari al 3,21 per cento del PIL. I dati dimostrano che, se il Paese vuole vincere questa battaglia (che è una battaglia di civiltà a difesa dell'incolumità e della salute sui luoghi di lavoro), occorre mantenere alta la tensione morale ed ideale. È una battaglia che tutti - Governo, Parlamento, istituzioni, forze politiche, forze sociali - si devono sentire impegnati a vincere. E questo ancor più adesso, in presenza cioè di una crisi economica che rischia di aggravare le condizioni di lavoro. Devo dire, a questo proposito, che Governo e Parlamento, partendo dalla legge delega 3 agosto 2007, proseguendo con l'approvazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e approvando per ultimo il decreto integrativo e correttivo 3 agosto 2009, n. 106, hanno messo in campo un imponente processo di riforma legislativa, tant'è che l'Italia può oggi contare su un complesso di norme e regole in linea con le migliori tradizioni europee ed internazionali. Impianto legislativo che, vorrei ricordare, è stato il frutto di un ampio confronto, e devo aggiungere, di amplissime condivisioni. Tessuto normativo, quello dell'impianto legislativo, per sua natura fortemente dinamico e che richiede, pertanto, periodiche manutenzioni e continui aggiornamenti. Manutenzioni ed aggiornamenti imposti, da un lato, dalla continua e tumultuosa evoluzione tecnologica e dal processo di innalzamento della cultura sociale in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; dall'altro, dall'impatto che il sistema normativo ha con gli ambienti di lavoro. Per quest'ultimo motivo il lavoro svolto sul campo dalla Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro può essere di aiuto e di supporto per il legislatore. Lavoro che quest'anno, così come quello approvato con la risoluzione dell'anno scorso, troverà una sintesi - mi auguro ancora unitaria - in una serie di proposte tese ad eliminare le criticità riscontrate a seguito di verifiche sul campo. Devo dire che a questo proposito mi sento di riprendere, in questa discussione, alcune criticità già evidenziate sia nella discussione che accompagnò l'approvazione della prima risoluzione della Commissione sia, ancor prima, nelle discussioni che accompagnarono l'approvazione del decreto legislativo n. 81 prima e del decreto correttivo n. 106 poi. Mi riferisco in particolare al sistema duale Stato-Regioni tuttora vigente in materia di vigilanza e controllo. È doveroso sottolineare, a tale proposito, che né il legislatore delegato del decreto legislativo n. 81 del 2008 (centrosinistra), né il legislatore delegato del decreto legislativo n. 106 del 2009 2009 (centrodestra) hanno avuto abbastanza coraggio per dare corso ad un superamento del sistema duale. Superamento, fra l'altro, previsto dalla legge delega n. 123 del 2007. Si sono mantenute, pertanto, in piedi le criticità tipiche di un sistema di vigilanza e controllo di tale tipo: sovrapposizioni, duplicazioni, carenze, vuoti nell'attività di vigilanza e controllo. Spero che Governo e Parlamento si facciano carico di tali disfunzioni e pervengano rapidamente ad un sistema unitario per ciò che attiene un settore importante quale quello del controllo e della vigilanza. Tralasciando per brevità e per economia di tempo altre criticità emerse nell'applicazione dell'impianto legislativo, fra l'altro evidenziate da chi mi ha preceduto, il dato più importante che va assolutamente sottolineato è che, a fronte di una positiva rivisitazione legislativa e normativa, non ha fatto riscontro, nella realtà quotidiana degli ambienti di lavoro e di produzione, quel cambiamento culturale da tutti auspicato ma che è ancora tutto da realizzare. La vera sfida che quindi oggi resta, ed è tutta da vincere, è quella di un cambiamento culturale radicale da parte di tutti i soggetti interessati, anche di fronte al banco di prova che è la crisi economica e che potrebbe indurre molte aziende - quelle più spericolate, quelle più spregiudicate, come è stato detto - ad intraprendere la scorciatoia dell'abbassamento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro per contenere i costi di produzione. Sfida per rafforzare essenzialmente gli strumenti culturali al centro dell'impianto legislativo vigente, quali la formazione e l'informazione. Solo elevando gli elementi di conoscenza di tutti gli attori in campo, lavoratori e datori di lavoro, attraverso la realizzazione di attività informative e formative, effettive ed efficaci, è infatti possibile elevare i livelli di tutela afferenti alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Solo attraverso attività formative effettive ed efficaci è possibile abbattere i rischi da lavoro, con particolare riferimento a quelli di tipo comportamentale, derivanti cioè da abitudini radicate nel tempo e responsabili della parte più consistente degli infortuni sul lavoro. Solo attraverso attività formative veramente effettive ed efficaci si può segnare, come dice il ministro Sacconi, una discontinuità rispetto ad un approccio meramente burocratico in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a favore di un approccio per obiettivi che implichi maggiore attenzione ai profili sostanziali piuttosto che a quelli formali. L'informazione e la formazione sono dunque elementi imprescindibili per un corretto approccio alla prevenzione. Bisogna però comprendere di quale informazione e formazione parliamo: della formazione strategica prevista nell'impianto legislativo o di quella al presente? L'impianto legislativo prevede, infatti, mettendo al centro la persona, una formazione e un'informazione riferita a ciascun lavoratore quale diritto individuale del lavoratore stesso. L'informazione e la formazione previste nell'impianto legislativo non sono, come si dice in gergo tecnico, un'obbligazione di mezzi, ossia un obbligo in testa al datore di lavoro per lo svolgimento di una certa attività (in questo caso l'erogazione dell'informazione e formazione indipendentemente dalla verifica in merito alla assimilazione da parte del lavoratore), bensì vanno inquadrate come un'obbligazione di risultato, ossia come l'obbligo di verificare l'effettiva assimilazione dei concetti e dei contenuti da parte dei destinatari della formazione e dell'informazione. Questa la formazione prevista nell'impianto legislativo, che può essere considerata a ragione una fondamentale leva strategica per l'affermazione di una cultura della prevenzione. Lontana anni luce dalla formazione strategica ipotizzata nell'impianto legislativo è la formazione presente, che, quando non elusiva, come avviene in molte realtà, viene vissuta come un obbligo un obbligo o un diritto - a seconda da quale parte lo si guardi - di natura formale cui adempiere in ossequio al dettato normativo. Si tratta in questi casi di formazione che si riduce alla consegna di opuscoli di contenuto del tutto generico o nella mera proiezione di *slide*, che ripropongono molto spesso il testo di legge. Si tratta di una formazione formale che non aiuta il paese nella lotta agli infortuni sul lavoro. Significativa a questo proposito sono le indagini

e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza attraverso la somministrazione di un questionario-intervista. Dalle risposte dirette dei lavoratori sono emerse forti criticità degli interventi formativi, necessariamente da affrontare e risolvere a livello organizzativo e di gestione aziendale in un'ottica di effettività. Su 1.000 intervistati, il 61 per cento dichiara di aver partecipato a corsi formativi, cento definisce non utile l'intervento formativo svolto; il 44 per cento ritiene che gli interventi formativi si siano limitati ad assolvere gli obblighi di legge per evitare le sanzioni. Il fatto che il 40 per cento dei lavoratori non abbia fatto formazione negli ultimi anni non è rassicurante e la dice lunga sul funzionamento dell'attuale sistema di formazione e sicurezza. Per quanto riguarda la cosiddetta formazione in ingresso, dall'indagine risulta che, a fronte di un 10 per cento degli intervistati che ha iniziato l'attività in affiancamento ad altri lavoratori e di una più bassa percentuale (6 che ha svolto veri e propri corsi professionalizzanti, la stragrande maggioranza dei lavoratori ha dichiarato che l'apprendimento del lavoro è avvenuto mediante esperienza maturata direttamente sui luoghi di lavoro. Il fatto che nella fase di ingresso soltanto il 10 per cento dei lavoratori sia stato affiancato implica e conferma, anzitutto, che la formazione in molti casi viene percepita solo come un obbligo di legge. Il dato è più preoccupante per i giovani e per i lavoratori atipici e non standard i quali avrebbero, più degli altri, bisogno di affiancamento. Sono dati che allarmano e che richiedono lo sforzo di tutti gli attori in campo assunte le responsabilità condivise introdotte per la prima volta dal decreto legislativo n. 106 del 2009per rendere effettiva la scelta compiuta dal legislatore tesa ad accrescere la cultura della prevenzione. coinvolgere tutti, a partire dal mondo della scuola che appare poco coinvolto pur essendo il luogo che dovrebbe essere, in via prioritaria, deputato a sviluppare fin dall'infanzia la cultura della prevenzione nei luoghi di vita prima e di lavoro poi. cultura della prevenzione e della sicurezza, come giustamente fa rilevare il ministro Sacconi, non dovrebbe essere trattata come materia separata ma come un valore pervasivo di tutte le materie scolastiche. A conclusione di questo mio breve intervento non mi resta che augurare buon lavoro a tutti

Commissione, il clima che vive la Commissione in riferimento ai temi sui quali è coinvolta e per i quali si interessa ed agisce.

riguardo il dibattito si è aperto sin da allora - il Ministro del lavoro è presente e ne è testimone - quindi credo che continueranno a coesistere sensibilità diverse su questo atto.

Probabilmente, anche nella sua replica, il Ministro farà riferimento a queste sinergie e a questa collaborazione su questo tema. Ecco, io inviterei i colleghi che hanno presentato le altre proposte di

che tutto ciò è stato legato alla definizione di un Regolamento. Quindi, questo ha richiesto tempo e, comunque, è in stato avanzato. Io sono convinto che il Ministro potrà confermare anche questo aspetto.

effettivamente lavorate. Quindi, vi sono elementi oggettivi, ma questo punto potrebbe essere sicuramente accolto. Così come potrebbe essere accolto, al punto successivo, la parte che è stata aggiunta e, più specificatamente, là dove si dice: «l'innovazione dell'assetto normativo preesistente e la sua riunificazione in un testo unico completo ed esaustivo quanto alla definizione di istituti, soggetti e funzioni del sistema della prevenzione e del contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro

contenendo la pratica del subappalto al fine di contrastare il deleterio fenomeno per cui l'abbattimento dei costi volto a garantire offerte più competitive si traduce spesso, da parte delle imprese più sleali e spregiudicate,

Presidente, desidero innanzi tutto esprimere un sincero apprezzamento per l'opera svolta dalla Commissione, non a caso conclusasi con una seconda relazione condivisa.

importante infatti che su un diritto vitale, come quello alla salute e alla sicurezza sul lavoro, si registri un'ampia condivisione, anche perché la materia, per la la regolazione istituzionale che vi presiede, implica forte concertazione tra istituzioni centrali e regionali ed amministrazioni, guidate guidate anche da maggioranze diverse, la cui collaborazione è assolutamente essenziale. Raccolgo, in particolare, un'osservazione svolta a tale proposito dal senatore Nerozzi, che condivido, circa la necessità di un'omogeneità su tutto il territorio nazionale. Come è noto, la riforma della Carta costituzionale, che poi non è stata confermata dal *referendum*, riportava nelle competenze centrali la materia della salute e della sicurezza sul lavoro. Mi auguro che un futuro lavoro condiviso a questo proposito possa condurre ad una scelta che consenta quell'omogeneità della disciplina, che è garanzia per la sua effettività, e quella di controllo, che certamente si realizza in termini ancora più efficaci se viene espressa da competenze unificate e non, come accade oggi, concorrenti.

ricordo come non solo si sia proceduto al coordinamento invocato dal Testo unico, ma come si sia in particolare provveduto ad integrare le capacità delle istituzioni centrali, in particolare quelle del Ministero del lavoro, con l'ausilio indispensabile dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Nello stesso tempo, la collaborazione operativa è necessaria soprattutto per contrastare le forme più odiose di sfruttamento del lavoro, quella irregolarità totale nella quale si produce un immanente pericolo per l'incolumità delle persone, come accade in un cantiere abusivo o in un opificio totalmente irregolare nel quale magari sono impiegati minori. L'attività di implementazione del Testo unico ha comportato processi non semplici per la volontà

di sollecitare concertazione con le parti sociali (la commissione consultiva ne è lo strumento fondamentale) e leale collaborazione con le Regioni. Questi percorsi concertativi, che sono in atto e che si articolano all'interno della commissione anche in numerosi gruppi di lavoro, sono talora ragione di lentezza nel processo di implementazione. È mia intenzione sollecitare le parti sociali a realizzare realizzare avvisi e posizioni comuni in termini molto più rapidi di quelli che si sono verificati ad ora. Tra le attività che sono in corso per il completamento normativo e per la dotazione di tutta la strumentazione che il Testo unico ipotizza, ricordo, in particolare,

di correggere quindi tempestivamente anche le azioni che conduciamo proprio in relazione ai risultati, che non possono essere considerati in termini aggregati date le fortissime diversità che si registrano nel nostro nel nostro tessuto produttivo e nel nostro mercato del lavoro. Questo sistema è stato ormai definito in termini informali tra le amministrazioni,

attività edili e, dall'altro, alla disciplina relativa agli ambienti confinati, posto che in essi abbiamo registrato una ripetizione una ripetizione di infortuni, anche con le stesse caratteristiche, nonostante l'attenzione degli organi di vigilanza dei servizi sanitari regionali. sanitari regionali. La patente in edilizia credo corrisponda all'impegno contenuto in alcune delle risoluzioni presentate a che si determini un filtro all'accesso ad un'attività professionale che risulta particolarmente esposta ai rischi per la salute dei lavoratori. La patente appare un modo per garantire competenze e conoscenze riferite alla salute e alla sicurezza coerenti con la disciplina comunitaria di accesso alle professioni. Per quanto riguarda invece gli ambienti confinati, il Governo è intenzionato, come già riferito alla Commissione, non soltanto ad accentuare le attività di

che ragionevolmente possono essere prodotti in sede di decretazione, quindi di regolazione secondaria, con riferimento, per esempio, alla presenza di un rappresentante dell'appaltante in tutte le attività degli appaltatori:

Per quanto riguarda le considerazioni svolte in materia di appalti, ricordo che la disciplina vigente appare, in teoria, completa e non consente compressione né dei costi del lavoro secondo i contratti collettivi, come rilevato dalle stesse tabelle prodotte in base alla cosiddetta legge Salvi dal Ministero del lavoro, né tanto meno dei costi relativi alla sicurezza.

pieno ottemperamento degli obblighi di legge, con riguardo al costo del lavoro e ai doverosi costi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in modo che la logica del massimo ribasso non possa in alcun modo comprimere comprimere questi obblighi fondamentali per l'impresa. Per quanto riguarda l'amianto, ringrazio il senatore Casson, che nella sua attività, professionale prima e parlamentare poi, ha sempre prestato molta e qualificata attenzione

il regolamento relativo al fondo per le vittime dell'amianto che, quindi, diventa operativo. Non è stato facile definire questo testo. Com'è noto, la materia ha dato luogo a molte ingiustizie, determinate talora da sottovalutazione

prodotto danni anche gravi alla salute, ma dall'altra parte abbiamo conosciuto anche molti abusi. Sono infatti in atto inchieste da parte di alcune procure per comportamenti che sono stati supposti come illegittimi da parte di aziende che hanno riconosciuto un certo grado di esposizione all'amianto in funzione di attività di prepensionamento dei lavoratori, con la conseguenza che si sono determinati negli stessi lavoratori diritti oggi difficilmente comprimibili, pur a seguito di comportamenti irresponsabili da parte dei datori di lavoro. Credo che dobbiamo evitare abusi e impropri riconoscimenti di Per quanto riguarda

cui ha parlato il senatore Roilo, condivido l'esigenza di fare qualcosa di più, e di farlo attraverso un'idea di presa in carico da parte dell'Istituto della persona che è risultata vittima di un infortunio o di una malattia professionale. Ciò, per fare sì che la presa in carico comporti un'assistenza alla persona lungo un intero processo, che deve realizzarsi realizzarsi anche con il reimpiego della persona stessa - al di là del grado di disabilità che può, in conseguenza dell'infortunio, aver - utilizzando l'INAIL stessa, in sussidiarietà, anche organizzazioni rappresentative, come l'Associazione appaiono in grado - proprio per la prossimità che le caratterizza rispetto alle persone - di svolgere una funzione utile al loro reimpiego, quale spesso

realizzato una positiva collaborazione tra le amministrazioni del lavoro e quelle dell'istruzione, ma ha anche coinvolto in sussidiarietà soggetti quali l'ANMIL.

soltanto con lo strumento sanzionatorio, che - come è stato prima osservato dal senatore Morra - talora dà luogo a comportamenti troppo formali, ad adempimenti di tipo formalistico.

se le parti sociali collaborano, ossia se il datore di lavoro e il lavoratore, le loro organizzazioni, collaborano, come spesso fanno, attraverso forme paritetiche ed enti bilaterali. La condivisione e la collaborazione costituiscono, infatti, un modo di adempiere ad alcuni requisiti formali in termini, però, sostanzialisti ci penso al modo con il quale si può redigere un documento di valutazione

corrispondere all'obiettivo della sicurezza non solo in termini formali. Questa, infatti, deve essere una preoccupazione comune. Sappiamo che, oltre una certa soglia, di fronte alla richiesta di un adempimento formale, il timore della sanzione può indurre a comportamenti formalistici che possono risolversi in una certa indifferenza rispetto all'effettività di un ambiente di lavoro sicuro. Possiamo evitare i rischi del formalismo solo se sviluppiamo le forme di condivisione fra organizzazioni dei lavoratori, degli imprenditori, datori di lavoro e lavoratori.

dirlo - al bene comune, al di là di differenze che possono muovere anche da approcci politico-culturali diversi ai rapporti di lavoro e alla loro ragione. Il Governo

volontà suprema dell'Aula, tanto più in una materia come questa.

e parimenti ad intervenire con opportune forme repressive nei confronti di quelle aziende che non ottemperano alla messa in sicurezza e/o sostituzione del macchinario obsoleto, che non

sebbene, come indicato nella seconda relazione annuale della Commissione d'inchiesta, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Italia abbiano mostrato negli ultimi anni un *trend* decrescente, segnale certamente positivo, i numeri restano tuttavia troppo elevati. Tra le varie concause che fanno dell'Italia un Paese in cui le morti sul lavoro sono ancora molte, la pratica del non assegnare - come invece previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - alle attività di prevenzione delle ASL le ingenti risorse provenienti dalle sanzioni incassate per le violazioni accertate. A peggiorare la situazione concorre la mancata attuazione di oltre 50 decreti attuativi del Testo unico, tra cui quelli che riguardano i rischi *stress*-lavoro correlati e la formazione di molte figure professionali della prevenzione: negli ultimi due anni l'85 per cento delle figure lavorative preposte non ha partecipato a veri corsi di aggiornamento sull'argomento. Tra le azioni da perseguire nella difficile situazione italiana, che vede la mancanza a tutt'oggi del 50 per cento degli operatori ASL incaricati delle attività di controllo e prevenzione mentre quelli che vanno in pensione non vengono sostituiti - la Commissione d'inchiesta si pone l'obiettivo di intervenire sulla lotta al lavoro nero e sommerso con un'opera di contrasto all'illegalità e di rafforzamento delle risorse da attuarsi a livello pubblico e professionale. Appare, quindi, indispensabile uno sforzo ulteriore, così come ci sembra la Commissione si stia proponendo, per cercare di prevenire e di contrastare il fenomeno, intervenendo su tre aspetti fondamentali: la formazione/informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull'applicazione delle norme ma anche l'introduzione di sanzioni deterrenti; il coordinamento fra tutti i soggetti sociali ed istituzionali competenti. In ambito formativo le risorse ci sono ma spesso si riducono solo a dei timbri che non corrispondono ad una reale formazione. Il rispetto degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere presunto, ma va accertato caso per caso in relazione a tutti i fattori mediante i quali va condotta la valutazione. Mi sembra anche giusto evidenziare come, così continuando ad operare, entreremmo, o meglio dire resteremmo, in contrasto con l'ordinamento comunitario che ha più volte ribadito l'orientamento secondo cui le semplici prassi amministrative non sono idonee a garantire l'esatto adempimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri. Perché ci sia sicurezza, oltre a prevenire è necessario anche controllare e sanzionare. In questo senso, mettere insieme tante associazioni nella Commissione d'inchiesta è un elemento importante perché è necessario unire le forze. Non a caso, l'altro filone di indagine del gruppo di lavoro è quello dei controlli pubblici in materia antinfortunistica, le cui competenze sono affidate ad una pluralità di organismi. In proposito, riscontro favorevolmente che la Commissione ha avuto modo di verificare, nel corso della sua inchiesta, l'esigenza di rafforzare in maniera sempre più incisiva il coordinamento e la collaborazione fra tutti gli enti istituzionali che si occupano, a vario titolo, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, Molte questioni sul tappeto sono state portate avanti dalla Commissione d'inchiesta, che ha svolto un lavoro veramente importante.

Tuttavia vi è un punto sul quale la proposta di risoluzione dell'Italia dei Valori concentra la sua attenzione: la richiesta, che abbiamo formulato anche in altre occasioni e che qui oggi reiteriamo, del ripristino del rigoroso sistema sanzionatorio previsto dal decreto n. 81 del 2008. Come sottolineato in tutte le proposte di risoluzione, in Italia ogni anno si continua a registrare un numero di infortuni e di morti sul lavoro che è inaccettabile in un Paese sviluppato. Non posso far altro che confermare qui la posizione che l'Italia dei Valori ha sempre espresso. È necessaria la valorizzazione del momento della prevenzione e della formazione del personale ma, insieme a ciò, è necessaria altresì altresì la predisposizione di un serio e rigoroso regime sanzionatorio, la cui effettiva applicazione deve essere garantita assicurando agli organi a ciò preposti l'assegnazione di congrue risorse sia strumentali che finanziarie ed umane. Non posso inoltre non registrare e condividere pienamente i rilievi sul tema della salute, sui luoghi di lavoro e sulla necessaria assistenza ai lavoratori colpiti da patologie di origine professionale, che ho potuto leggere nella proposta di risoluzione dei colleghi del Partito Democratico. Concludo, signora Presidente, annunciando il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori, ovviamente alla nostra proposta, a prima firma della senatrice Bugnano, ma anche alla proposta di risoluzione n. 2, a prima firma del e l'astensione del nostro Gruppo sulla proposta di risoluzione n. 1, a firma del presidente Tofani, perché manca un riferimento incisivo al sistema sanzionatorio che per noi - ripeto - è prioritario

Purtroppo, il sistema complessivo di prevenzione e sanzione non funziona; siamo di fronte a morti continue: quattro soltanto ieri, un'ultima stamattina, signor Presidente, un altro morto nel Salento, qualche ora fa. Dobbiamo davvero mettere fine a questa carneficina. Come Italia dei Valori, ci impegneremo a lavorare all'interno della Commissione per raggiungere una posizione il più possibile condivisa sul sistema delle sanzioni perché - ripeto - la tutela del lavoratore è un punto fondamentale, come ultimamente ci ricorda molto spesso anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano.

Esprimo altresì un giudizio positivo sulle proposte di risoluzione dell'opposizione, sicuramente apportando le modifiche già illustrate dal presidente Tofani, visto che comunque - volevo ricordarlo soprattutto ai colleghi che

La seduta è tolta